Se ho ben capito, il senatore Polledri, oltre a chiedere la verifica del numero legale, ha posto anche il problema del voto sul processo verbale. Anche se non ha chiesto aggiustamenti o ritocchi specifici, ha parlato di un processo verbale che non dà il senso

Grazie,

Signor Presidente, nessuno voleva scomodare la letteratura italiana, solo che mi sembrava di non aver ben colto

Lei ieri ha usato una grande cortesia nei miei confronti: ha fatto rispondere il presidente Angius su una questione delicatissima, legata all'esame di un provvedimento che viene approvato sotto la forma del decreto-legge e alla fattispecie, prevista per il Senato e non per la Camera, nella sua procedura dall'articolo 78 del nostro Regolamento sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Dico subito in premessa che non è mio costume mettere in discussione una decisione del Presidente del Senato perché credo che, se vi è un elemento di garanzia in Aula, esso è rappresentato dalla Presidenza. Quindi, posta una questione e ricevuta una risposta, credo che l'Assemblea debba tenerne conto e vale ovviamente anche per il futuro. C'è una carenza - ho letto con attenzione la nota preparata e poi sostenuta in Aula dal presidente Angius - che stabilisce sostanzialmente, anche alla luce dell'intervento della presidente Finocchiaro nel dibattito, che resiste il principio stabilito dall'articolo 78, per cui ciascun senatore può chiedere che un articolo, un comma, una frase

se non vi sono osservazioni, è pacifico che il Presidente possa decidere di andare avanti, ma se il Presidente ha dubbi fa votare per alzata di mano senza discussione. Non ne sono convinto, ma accetto la decisione della Presidenza: non si può fare altrimenti perché sarebbe irrispettoso e irriguardoso delle nostre regole. Accetto che l'articolo 78 del Regolamento venga fatto sopravvivere, più che vivere,

che venga posta in votazione la parte separata di un provvedimento vale, ad esempio, la fattispecie prevista dall'articolo 89,

si rischia di non trovare la sopravvivenza del principio stabilito dall'articolo 78 del Regolamento né in Commissione né in Aula. Credo che su questo diritto di motivazione debba essere data una certezza da parte del Presidente, posto che - pur non condividendole - si accettano le decisioni della Presidenza.

la possibilità di motivare la richiesta di votazione per parti separate e addirittura la possibilità di dichiarazione di voto. I precedenti del 2006 sono, sotto questo profilo, negativi visto che non è stato consentito al senatore Saporito

Il precedente del 1994, che vedeva protagonisti i senatori Ronchi e Salvi, è in linea assolutamente difforme,

e al senatore La Loggia di procedere alla dichiarazione di voto, come da resoconto stenografico. Quindi, i precedenti sono tra loro contrastanti in ordine alla corretta interpretazione del Regolamento. Ilsecondo punto riguarda

si è stabilito che, in caso di più richieste di votazioni per parti separate, la decisione in ordine a tali richieste sarebbe avvenuta con un'unica votazione sarebbe avvenuta con un'unica votazione per alzata di mano, adducendo a sostegno di questa affermazione la presenza di precedenti e, in particolare, in sede di Commissione di quelli del 2006. 2006. Presidente, non voglio dire che l'articolo 102 del Regolamento fa riferimento alla votazione degli articoli e degli emendamenti, perché già questo, per la verità, potrebbe essere un buon argomento da spendere. che accedere a una votazione complessiva evidentemente comporterebbe, se uno volesse votare favorevolmente solo a una delle proposte, votare favorevolmente a tutte le proposte, anche a quelle che non si condividono,

per parti separate tutti i singoli articoli e di una richiesta di votare per parti separate solo ed esclusivamente l'articolo 1,

Presidente, sinceramente mi dispiace che l'Aula debba frequentemente occuparsi delle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione che ho l'onore di presiedere. Trovo personalmente anche abbastanza irrituale che ciò avvenga; se dovesse avvenire per tutte le Commissioni credo che i lavori dell'Aula verrebbero interamente dedicati a tale questione,

Per quanto riguarda la questione sollevata, ho inteso ritenere che le modalità di esame da parte della Commissione affari costituzionali dei presupposti di legittimità ed urgenza rispondessero a una particolare necessità e cioè che la Commissione ha il dovere di esprimere il suo parere sull'esistenza dei presupposti e di farlo in un tempo ragionevole. Ho ritenuto che, in assenza di specifiche previsioni per i lavori della Commissione, valessero i princìpi e le norme procedurali previste per i lavori dell'Aula. Sono stato confortato in tale decisione dal suo orientamento e naturalmente accetto con grande piacere, com'è ovvio e naturale, che la Giunta per il Regolamento esamini ulteriormente la questione e dia un definitivo parere. Voglio però informarla, signor Presidente, che ieri sera, nonostante l'avviso che ella ha autorevolmente fornito, la Commissione - era la quarta seduta in cui ci occupavamo della questione relativa ai presupposti sul decreto in oggetto in oggetto - ha egualmente proceduto a votazioni per parti separate, dato che nessuno dei membri della Commissione aveva sollevato alcuna questione. Non vi è stato neanche il bisogno di procedere a votazione per ammetterla. Le dico di più, Presidente: a differenza di quello che è stato detto, è stata data la parola ai colleghi che l'hanno richiesta per illustrare la richiesta di votazione per parti separate, tant'è vero che ci sono state quattro votazioni per parti separate e poi la votazione definitiva.

che è stata comunicata dal presidente Angius ieri nel corso della seduta dell'Assemblea, è una nota, a mio avviso ovviamente, corretta nel merito e nel modo in cui è stata proposta.

Io avrei potuto esprimere il nostro orientamento, l'interpretazione, sulla base anche di precedenti discutibili (il senatore Palma, ad esempio, ne ha trovati altri che rimettono in discussione la questione), ma avevamo anticipato questo rischio e, per il rilievo della questione posta, abbiamo affidato a due senatori la preparazione dell'istruttoria per questo e per qualche altro problema che l'Aula, nel corso di queste ultime settimane e mesi ha posto. Arriveremo ad un chiarimento nella Giunta su questa faccenda. faccenda. Vi ringrazio anche per il modo serio con cui questo problema non trascurabile è stato posto all'attenzione dell'Aula. ai banchi della maggioranza)* Io però non accetto questo ricorso al coro quando il Presidente si sta rivolgendo a un senatore che chiede qualcosa. No, senatore Storace, mi pare che ulteriori domande

risiede anche la possibilità, in una certa situazione, di consentire comunque l'illustrazione della richiesta, anche sulle questioni procedurali. Su quel punto il Regolamento recita: «senza discussione». Cosa impedisce al Presidente

e una legge del Parlamento italiano, precisamente la legge 15 aprile 2005, n. 61, nel suo «La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre "Giorno della libertà", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo».

e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti». Io credo che sede più alta non possa esserci, per ricordare questa data; mi posso solo rammaricare che il Governo non abbia preso l'iniziativa di farlo. La data è in ricordo del «Giorno della libertà»;

essenzialmente nell'ambito dei problemi europei e, in modo particolare, di quelli della Germania federale (ho scritto anche un libro su Brandt e sulla *Ostpolitik*, che potrei citare, ma naturalmente questa sarebbe un'auto-*reclame*): la caduta del muro di Berlino, il suo abbattimento fisico voleva significare l'abbattimento del comunismo, vale a dire di quel sistema che aveva impedito non solo la riunificazione della Germania (per la quale d'altra parte esisteva anche qualche dubbio), ma di un regime che aveva oppresso. La forza per abbattere il muro di Berlino fu scatenata dalla rivoluzione ungherese; fu scatenata dalla opposizione all'occupazione della Cecoslovacchia: fu questo un moto che dal popolo dell'Est europeo si manifestò.

di ricordo di questa giornata come ricordo dell'abbattimento di un sistema comunista che ha oppresso per molti anni l'Est europeo e dal quale, col voto libero di questi cittadini, l'Est europeo si è liberato.

Commissione, che prego il senatore segretario di voler leggere. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.2 (testo 2) e 5.303 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

vorrei semplicemente far osservare che la proposta di modifica 5.2 (testo 2) che è sostanziale, doveva recare la firma o del Governo o del relatore, non essendo passata attraverso la Commissione. È una modifica talmente sostanziale che aveva bisogno di un paternità chiara; il relatore ha ritenuto di doverla attribuire all'intera Commissione, ma la discussione in Commissione non vi è stata. Per dovere di procedura, devo assolutamente significare

a firma dei Capigruppo in Commissione ambiente di tutti i Gruppi della Casa delle Libertà, vive, in quanto agganciabile anche al testo nuovo della Commissione. Ripeto: sul merito delle due proposte (il nostro subemendamento

Presidente, l'osservazione del senatore D'Alì, da un punto di vista formale, è corretta, anche se l'emendamento 5.2 (testo 2) è frutto della discussione svoltasi in Aula e precedentemente in Commissione, raccogliendo gli emendamenti presentati in entrambe le sedi, in particolare dal senatore Palumbo e dal senatore Barbato e con l'integrazione del senatore Morra.

Presidente, può rileggerci la riformulazione del testo, visto che non tutti la conoscono? c'è uno stampato che è stato distribuito.

le osservazioni del senatore Libé, le condivido e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione. Ritengo che, rispetto al testo del decreto originario, facciamo notevoli passi avanti. Voglio ricordare che erano già previste nel decreto le discariche, discariche

in più aggiungiamo un elemento che non riguarda solo quelle due discariche: disponiamo che, nell'individuazione delle aree, il commissario dovrà tener conto anche degli impatti ambientali gravanti per passati utilizzi di quei territori. Credo che ci sia

il massimo che possiamo fare, in considerazione del fatto che comunque stiamo dando poteri straordinari a un commissario per fronteggiare una situazione di emergenza, quindi è evidente che alcune deroghe verranno fatte.

svolto in Commissione, il quale ha perfezionato *in* *toto* il provvedimento, penso non sia poi così difficile sostituire, tener conto ed escludere: non cambia la sostanza dell'intendimento che la Commissione ha voluto dare a quel provvedimento.

di una tutela per i territori che hanno discariche esaurite e non ancora messe in sicurezza per mancanza di risorse. Si individua anche un percorso per dare priorità alla messa in sicurezza delle discariche esaurite.

Presidente, può darsi che io sia in errore e le chiedo pertanto di aiutarmi a fare chiarezza. Guardando il testo degli emendamenti, vorrei sapere, perché nella confusione non sono riuscito a comprenderlo (quindi sarà una mia colpa), che fine ha fatto l'emendamento 5.303

dell'emendamento 5.300, ma la richiesta del senatore Ronchi era relativa alle modifiche proposte dal senatore Libé al comma 3,

il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione. Può, quindi, sospenderlo, senza sentire, intendere o concertare con nessuno.

rifiuti i presidenti delle Regioni non contano nulla e rimandiamo i rifiuti a casa senza nessuna possibilità di dibattere. Ebbene, ritengo che il «sentiti» sia troppo debole non vogliamo scrivere «di concerto» almeno dobbiamo scrivere «d'intesa» perché altrimenti si crea all'interno di questo provvedimento una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile e i poteri del commissario diventano addirittura superiori di quelli dei presidenti delle Regioni. Questo mi pare che non possa essere assolutamente accettato. temo che il senatore Matteoli abbia messo insieme due materie differenti. La questione del commissario, che può impedire l'ingresso, riguarda i rifiuti speciali; la trasmissione di rifiuti fuori Regione si riferisce a rifiuti solidi urbani, i quali, per legge, non possono essere trasferiti fuori Regione. Allora, si tratta di due questioni completamente differenti. Si tratta di decidere se il commissario deve andare in altre Regioni. Quello del senatore Morra è ancora un altro emendamento: si riferisce alla realizzazione di discariche in prossimità della zona di confine, per le quali si chiede

responsabile del territorio pugliese dirà: «Per cortesia, se ci vogliamo sentire prima di fare altre cose di questo genere è meglio». Si tratta, quindi, di tre fattispecie del tutto differenti:

a questo, siccome si sa che la situazione in alcuni territori della Campania è totalmente fuori controllo, si vuole mettere si vuole mettere una pezza ad una condizione paradossale per cui la Campania, che non ha capacità di smaltire i suoi rifiuti, poi accoglie migliaia di tonnellate di rifiuti speciali da altre Regioni, spesso fuori da ogni controllo concreto di tranquillità sul trattamento dal punto di vista ambientale. Quindi, quantomeno che siano chiare le tre fattispecie differenti sulle quali si interviene in maniera, a nostro parere, non contraddittoria. il senatore Piglionica dice delle cose evidenti. Però prendiamo il provvedimento. Alla fine del nostro dibattito ci sarà il voto; se passerà questo provvedimento ci saranno tre trattamenti diversi, mi rendo conto, su specifiche di rifiuti diversi, ma con atteggiamenti completamente diversi; chiedo, quindi, che almeno il commissario sia parificato ai presidenti delle Regioni, che vengono eletti, affinché ci sia un comportamento uguale tra un presidente della Regione e il commissario.

Oggi i giornali pubblicano interventi di esponenti politici di tutte le Regioni d'Italia - di destra, di sinistra e di centro - che dicono: «Basta, non vogliamo più rifiuti della Campania da nessuna parte».

per consentire che il commissario possa concordare con il presidente della Regione, altrimenti i rifiuti resteranno in Campania perché nessuno li farà uscire.

specialmente a Napoli e in Campania, che i commissariamenti vengono spesso utilizzati come occasione per deresponsabilizzare le autorità locali e scaricare sul commissario responsabilità che invece vanno condivise, coinvolgendo in operazioni così delicate le opinioni pubbliche e i cittadini, che le autorità locali più di altri rappresentano. Troppe volte a Napoli e in Campania è accaduto che problemi ordinari, riguardanti l'economia e la società, siano stati capziosamente trasformati in emergenze, per scaricarli sui prefetti e sui questori, sollevando le autorità locali dalle loro responsabilità ma, al tempo stesso, dequalificando e squalificando i poteri locali. Allora, onorevoli colleghi, lasciamo stare, su questo punto,

Non c'è un limite, non c'è un'indicazione precisa, non c'è quel coinvolgimento al quale faceva riferimento il senatore Pisanu. Non solo, ci sono zone, come il giulianese, l'aversano, il paretano, che sono invase, ammorbate, avvelenate da decine e decine di discariche.

Anche le cose importanti che dice il senatore Pisanu c'entrano poco con l'emendamento che stiamo discutendo. È un discorso in generale, che abbiamo svolto nella discussione generale di ieri e che riprenderemo durante le dichiarazioni di voto, ma non ho capito, anche a proposito delle osservazioni del senatore Giuliano, a quale emendamento si riferiscano. Noi stiamo parlando di altre cose.

l'emendamento 5.8 non è ritirato: c'è stato un errore. Infatti ho chiesto al relatore di esprimere il parere

Presidente Sodano, ho qualche difficoltà a capire il testo che uscirà da questa seduta del Senato, perché la collega De Petris presenta un emendamento condivisibile, per carità, ma che va oltre. Qui si chiede addirittura il coinvolgimento degli enti locali: benissimo, ma allora come si fa a dire di no

il relatore Sodano ha detto una cosa diversa da quella che lei sostiene: ha detto di inserire su tutti e tre i problemi che ho sollevato la parola «sentite». Non sono d'accordo e chiedo che sia scritta, a proposito dei tre problemi che ho sollevato, le parole «d'intesa».

Presidente, ho formulato l'emendamento 5.11 alla luce della originaria impostazione del decreto, ma soprattutto per segnalare la titolarità dell'area su cui insiste da anni la discarica "Difesa grande"**,** che non è di proprietà del Comune e che necessita un intervento per evitare che si continui a determinare una condizione per cui vi è un peso pubblico e un interesse e un ricavo privato nella gestione dei rifiuti. In termini di moralizzazione, ho voluto segnalare un dato, un problema, nella consapevolezza che l'emendamento non ha copertura finanziaria. Sono il primo a saperlo. Era una provocazione ed una riflessione

un maggiore e tempestivo intervento delle forze dell'ordine nel caso in cui gli abitanti della Regione continuano ad adottare quei comportamenti di cui siamo stati buoni testimoni nella passata legislatura. Abbiamo visto poche centinaia di persone bloccare Via del Corso e gli accessi proprio per un problema legato ai termovalorizzatori e alle discariche. Chiediamo l'approvazione di questo emendamento per garantire ed accelerare gli interventi delle forze dell'ordine a difesa

Grazie,

passiamo al voto

Presidente, l'emendamento 5.120/2 vuole mantenere le dotazioni finanziarie nei limiti del programma. Non vorremmo disturbare il commissario, ma neanche il presidente Bassolino e portargli via una lira. Il presidente Bassolino è impegnato in cose più importanti dei rifiuti. Ricordo

sarebbe quello di eliminare il limite alle dotazioni finanziarie del POR della Regione Campania. L'emendamento in esame mobilita le risorse della Regione, ovviamente nei limiti di quelle esistenti.

parere favorevole

voglio sottolineare, anche per chi ci ascolta, che questo tono da stadio è assolutamente inaccettabile. Se si ripete, tolgo la seduta. Le urla no.

il seguente:* «2-*bis.* Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento

Presidente, io avevo svolto un intervento su tre emendamenti. *(Vivaci

sull'emendamento 5.303 (testo 2), ha la parola il senatore Matteoli. MATTEOLI *(AN)*. Credevo di non poter parlare. Noi abbiamo votato due precedenti emendamenti partendo dal presupposto che

*(Ulivo)*. Il senatore Matteoli, che ha svolto per cinque anni il delicatissimo compito di Ministro dell'ambiente e che ha dovuto quindi, anche in quella occasione, affrontare grandi emergenze, può immaginare quale complessità si avrebbe se, quando si va vicino ad un confine, ci si deve mettere nelle condizioni di raggiungere l'intesa con l'altra Regione? Si rischierebbe di paralizzare l'azione di un commissario che abbiamo istituito come tale perché avesse possibilità d'intervento un po' fuori dall'ordinario. Non si può trasformare tutto in un elemento di paralisi.

l'attenzione del Senato, in particolare dei colleghi della maggioranza, sulla questione or ora risollevata dal collega Matteoli. Per essere chiari, non siamo di fronte soltanto ad un problema, pur importantissimo, di carattere ecologico: siamo dinanzi ad un delicatissimo problema di sicurezza e di ordine pubblico che non può essere gestito senza una reale partecipazione delle autorità locali e delle popolazioni locali. Per intenderci, esemplificando, signor Presidente, a noi è accaduto qualche anno addietro che, per aprire ad Acerra il cantiere per il termoconvertitore, abbiamo dovuto mobilitare 1.000 uomini della polizia e contemporaneamente ci siamo trovati col commissario e la polizia da un lato e dall'altro lato gli amministratori comunali di Acerra, la popolazione locale e - in non gradita e certo occasionale compagnia - i camorristi gestori del ciclo dell'immondizia. Il problema è di evitare che situazioni sciagurate come questa abbiano a ripetersi; l'esigenza è di raccordare efficacemente, nella difesa di obiettivi comuni di ordine pubblico e di sviluppo, commissario, autorità locali e popolazioni locali. Questo è il problema reale e non possiamo eluderlo, colleghi, con giochetti di parole. Presidente, al di là delle riflessioni e delle considerazioni di ordine generale, l'emendamento esprime una realtà che già ha avuto modo di manifestarsi, che nasce da un'esigenza reale, che richiama alla complessiva responsabilità istituzionale, perché altrimenti si verifica il paradosso di una scelta necessaria e di un gioco delle parti tra presidenti delle Regioni, com'è accaduto esattamente per l'emendamento cui fa riferimento il senatore Morra: scelte necessitate in Campania, con la Puglia che invece organizza la contestazione perché non vuole la discarica a ridosso del confine con la Regione Puglia. Questo emendamento serve a determinare una condizione di responsabilità e di corresponsabilità istituzionale e rende la vicenda rifiuti non una vicenda localistica, ma di responsabilità dell'intero sistema. Presidente, noi dobbiamo fare uno sforzo, lo dico soprattutto ai colleghi dei Gruppi dell'opposizione, per evitare di sovrapporre fra loro molte fattispecie. Al senatore Pisanu, se me lo consente, desidero dire che è stata preoccupazione costante, nel corso dell'esame in Commissione, quella di evidenziare tutte le possibili associazioni di corresponsabilità di tutti i livelli istituzionali interessati alle scelte difficili del commissario. Siamo quindi pienamente d'accordo per quanto riguarda questo Dopodiché, sono nati tre problemi delicati: uno è quello della continuazione dell'arrivo in Campania dei rifiuti speciali da altre Regioni, e lo abbiamo risolto dicendo che il commissario può disporre la sospensione dell'arrivo di questi rifiuti speciali in Campania, salvo che non si faccia un esame supplementare; è nato poi il problema delle discariche che si possono collocare in zona di confine, e qui, per sovrappiù, anche rispetto all'esperienza passata, abbiamo identificato la possibilità

dei rifiuti dalla Campania ad altre Regioni, e qui abbiamo accettato la riformulazione che prevede l'intesa con la Regione ricevente. Credo che tutta la materia abbia trovato una sistemazione ormai equilibrata, anche dal punto di vista istituzionale. Mi rendo conto della delicatezza della materia, ma anche della necessità di una operatività in stato di emergenza. essa non viene assicurata, è inutile aver nominato il commissario ed è inutile aver designato a tale funzione il Capo del Dipartimento della protezione civile.

penalizzate e in qualche caso anche azzerate. Ecco perché, alla luce di questi dati, mi sembra utile e opportuna l'interpretazione del presidente Sodano. vorrei solo sottolineare, anche in risposta all'intervento del collega che mi ha preceduto, che questa non è una norma di carattere generale, ma riguarda soltanto la fase emergenziale, cioè una fase gestita con i poteri commissariali. Mi meraviglio come certe sensibilità non vengano raccolte, specialmente dai banchi della maggioranza, sempre molto attenta a che le emergenze di qualsiasi natura non si scarichino sui deboli. Qui si tratta di esperienza vissuta, quella della Puglia al confine con la Campania che sta sopportando quasi per intero l'emergenza campana. Si tratta, infatti, di un territorio debole, dove è più facile gestire la protesta sociale.

l'obbligo di sentire la Regione confinante. Ma non dobbiamo mettere il presidente della Regione confinante in un rapporto di sudditanza nei confronti del commissario.

di residui e di immondizie ad altre Regioni, debbano vedere coinvolti i Consigli regionali e non solamente, come genericamente

Passiamo all'emendamento 5.0.2,

Un divieto assoluto di gestire qualsiasi tipo di rifiuto speciale proveniente da altre Regioni potrebbe costituire un serio ostacolo

e che, quindi, utilizzano scarti di produzione e prodotti di rifiuto derivanti da altri che giungono in Regione Campania. L'emendamento della Commissione è differente, in quanto consente al commissario delegato la facoltà di verificare e regolare

mette il commissario stesso nella condizione di diventare una sorta di soggetto che fa assistenza tecnica alla Regione Campania, perché propone le modifiche del piano cave. Il commissario dispone le modifiche del piano cave, non le propone al presidente della Regione; non possiamo determinare una condizione tale per cui nella Regione Campania c'è il commissariamento dei rifiuti e la Regione vuole continuare a gestire alcuni ambiti e alcuni settori. Allora, si assuma la responsabilità complessiva il presidente della Regione e faccia anche il commissario straordinario di Governo per i rifiuti; altrimenti, prenda atto del fallimento complessivo e metta il commissario nelle condizioni di procedere rispetto alle omissioni della Regione anche per il piano cave.

Quindi, siccome chi oggi ha poteri straordinari per aprire nuove discariche o nuovi siti di stoccaggio, o per impedire che ciò avvenga a ridosso di aree già

pensiamo che con l'emendamento 5.260 si intervenga per introdurre un elemento di tutela per quei territori che sono già penalizzati dalla presenza di attività estrattive, per poterne limitare comunque l'attività. alcuni casi, di cui abbiamo discusso a lungo stamattina ed anche ieri, come quelli di Tufino e Ariano, sono a ridosso di cave che hanno divorato intere montagne. In quei casi è una forma di tutela; ritengo

il fatto che ci sia qualcuno che continua a fare il commissario per le cave e non vuole fare il commissario per i rifiuti, mentre quest'ultimo ha difficoltà operative e deve interfacciarsi con chi resta a fare il detentore del potere in relazione alle cave, rallenta il processo di tutela e di operatività. Allora, troviamo un meccanismo che recuperi meglio lo spirito. Comprendo perfettamente

diciamo «dispone d'intesa» o «determina d'intesa». Non è possibile però che di fatto ci sia un blocco da parte di chi ha assunto una posizione di deresponsabilizzazione rispetto alla vicenda rifiuti; un potere di blocco e di veto

Le argomentazioni del senatore Viespoli sono assolutamente opportune. A me pare che l'emendamento 5.260, tra l'altro, si presti anche ad un'evasione della normativa ordinaria sulle cave, attraverso la possibilità di una modifica a regime. Credo pertanto che si potrebbe trovare una soluzione,

Presidente, credo che siamo arrivati al punto fondamentale della discussione. Abbiamo giustamente analizzato, con approfondimenti utili, i poteri del commissario e i suoi raccordi con le istituzioni sul territorio,

da momenti purtroppo stabilizzati nel corso dei precedenti commissariamenti, uno dei quali è certamente l'assunzione, nei primi mesi dell'anno 2001, di ben 2.314 LSU a tempo indeterminato, assunzione che fa gravare sui conti della gestione commissariale importi per circa 55 milioni di euro annui. Allora, se il decreto non dota adeguatamente la gestione commissariale di risorse, insieme ai poteri di massima e pubblica sicurezza che stiamo dando al commissario straordinario dovremmo dargli anche quello

dovrebbe essere in grado di quantificare le esigenze di spesa di un commissariamento straordinario, anche sulla base di un'esperienza maturata nell'arco di un decennio ed oltre. Questa è la prima censura che muoviamo: allora, non avendo una relazione tecnica del Governo su tale previsione di spesa, non possiamo consentire che la copertura del decreto sia indeterminata nella sostanza e soprattutto nelle fonti, perché il rischio vero di questo decreto, così come articolato, è che le fonti di finanziamento della gestione commissariale ancora una volta ricadano sulla popolazione campana

consona alla realtà del nostro ordinamento fiscale di quanto non prevedesse il Governo o non avesse previsto la Commissione in prima battuta; abbiamo cioè eliminato quella dizione assolutamente atipica della tassa di smaltimento della Regione campana: tassa che non esiste nell'ordinamento e che se fosse stata mantenuta nel testo poteva anche suscitare la fantasia fiscale di questo Governo come nuova forma di imposizione, e sappiamo quanto pericolosa sia la fantasia fiscale di questo Governo in tema di vecchie e nuove tasse.

chiarisse che la TARSU non subisce e non può subire, per opera della gestione commissariale e neanche nel periodo della gestione commissariale, variazioni in aumento. Diversamente, se abbiamo risolto il problema formale dell'inquadramento di una fonte fiscale esistente, non abbiamo risolto il problema sostanziale della possibilità di aumento a danno dei cittadini campani di quella di quella imposta. Quindi, intanto questo sarebbe assolutamente indispensabile. In secondo luogo, sarebbe molto meglio evitare il riferimento a qualsiasi forma di imposizione che - ripeto - lascia libera la possibilità dell'aumento delle stesse imposte, con un riferimento preciso all'individuazione da parte del Governo di una somma congrua. Sappiamo bene che anche gli 80 milioni di euro che proponiamo non saranno sufficienti per l'intero periodo di attività, ma sappiamo bene che già per effetto dei meccanismi esistenti, il commissario può utilizzare i proventi TARSU dei Comuni che non provvedono direttamente al servizio e possono quindi riversare nella gestione commissariale le somme destinate a quel servizio. Ma c'è di più. Nella formulazione della Commissione i 20 milioni del 2006, che teoricamente potrebbero essere sufficienti a coprire questo mese e mezzo di periodo commissariale del 2006, sono per spese in conto capitale, mentre abbiamo un carico di spese correnti di 55 milioni l'anno, relativi agli LSU assunti nei primi mesi del 2001, guarda caso prima delle elezioni politiche, dal commissario Bassolino. Allora, questo carico

che la Commissione, su suggerimento del Governo (anche lì ho fatto le mie eccezioni procedurali ad inizio di seduta), ha inserito nel nuovo testo della Commissione, non sono assolutamente disponibili per spese correnti e quindi metteranno il commissario straordinario nelle condizioni di non poter pagare gli stipendi del personale a suo tempo assunto dalla precedente gestione commissariale. In più, avendo indicato solamente 20 milioni per il 2006, si rimane alla mercé della prossima legge finanziaria o di qualsiasi altro eventuale provvedimento ancor più tardivo, e quindi ancor peggio più tardivo, per determinare le risorse per il 2007. Non ci siamo.

l'emendamento della Commissione, sarà indispensabile approvare l'emendamento 5.0.1, che prevede un meccanismo di cartolarizzazione delle risorse dei Comuni attraverso i contributi erariali erogati dal Ministero dell'interno, in maniera tale che il commissario abbia certezza di fondi per la gestione commissariale. L'emendamento 5.0.1,

con riferimento a tale detto, abbiamo sempre, come Parlamento, autorizzato la deroga al Patto di stabilità medesimo per gli effetti delle spese dei Comuni in ordine alle gestioni commissariali.

si è sempre pronunciata contro questi interventi da parte dello Stato per due motivi sostanziali. Il primo riguarda una questione di giustizia nei confronti di tutti i cittadini italiani. Voglio ricordare che tutte le Regioni italiane

risorse non disponibili e ovviamente, trattandosi del disegno di legge finanziaria, ancora da approvare. Capisco la necessità di mettere una bandiera, però qui non c'è un'effettiva copertura e quindi non c'è alcuna disponibilità aggiuntiva. Il testo che stiamo approvando ha cercato invece di affrontare un problema che riguarda certamente la Campania ma che è di portata generale - la ragione per cui si ricorre a un commissariamento abbiamo risolto la questione della tariffa regionale, come emerso dal dibattito, precisando la destinazione della TARSU. Credo che non si possa bloccare la TARSU per legge, perché tale tassa riflette determinati criteri fissati per legge e quindi quella è. Sono state individuate risorse aggiuntive a supporto della raccolta differenziata con i contributi del CONAI. Anche qui non si tratta di un atto non dovuto perché il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi)

Infine, per i due mesi restanti si mobilitano 20 milioni di euro. C'è un ordine del giorno della Commissione, perché siamo in sessione di bilancio e ovviamente vogliamo impegnare il Governo

delle misure di emergenza, avendo però già indicato il fondo speciale per la Protezione civile. Penso quindi che l'emendamento 5.100/1

Presidente, stiamo esaminando un provvedimento molto importante, la discussione del resto lo evidenza. Ritengo che lei abbia scelto saggiamente di permettere anche ai Gruppi che hanno terminato il loro tempo di poter intervenire, proprio perché i temi che affrontiamo sono importanti. Tuttavia, signor Presidente, il suo invito alla stringatezza deve essere fatto rispettare. Se ci sono Gruppi che hanno terminato il tempo e che hanno esigenza di fare dichiarazioni di voto

delle dichiarazioni di voto finali i tempi verranno rispettati. Del resto, il livello e anche la capacità di risolvere qualche problema in Aula nel dibattito serrato che si è svolto questa mattina non è cosa che ricorra spessissimo nei nostri lavori. C'è stato un dibattito sereno e costruttivo ed alcuni problemi sono stati risolti, comunque ho presente il suo richiamo.

Presidente, avevo chiesto al relatore se non intendesse aggiungere, dopo la parola «TARSU», le parole: «per come oggi determinata e senza possibilità di incrementi». Quindi volevo avere una risposta in ordine a ciò. Il senatore Libé aveva inoltre chiesto se lei non intendesse mettere ai voti la parte finale dell'emendamento 5.300, che nella votazione per parti separate era stato accantonato sino alla discussione del comma 6 dell'articolo 5. Su questo chiedo che anche l'Aula possa essere informata.

Presidente, io credo che non sia accoglibile la sollecitazione del senatore D'Alì, perché noi non possiamo intervenire: la TARSU è la tariffa che applicano i Comuni; con i poteri commissariali interveniamo sulle

per il conferimento dei rifiuti e i Comuni pagano per il conferimento dei rifiuti oggi presso il CTR e domani presso le discariche, una tariffa che è applicata sulla base di un calcolo dei costi, non stiamo determinando dei costi aggiuntivi. Le risorse, come spiegava il senatore, Ronchi, ci sono. Del resto, questo decreto interviene per sostituire il prefetto Catenacci, che era stato nominato con un precedente decreto e quindi una parte delle risorse sono già disponibili presso il commissariato, perché è cambiato solo il commissario, da Catenacci a Bertolaso. Qui troviamo 20 milioni in aggiunta perché c'è una nuova situazione d'emergenza, determinata da quei 5 milioni di tonnellate di rifiuti. Per quelle riteniamo che per due mesi bastino i 20 milioni di euro, con l'ordine del giorno aggiuntivo, che voteremo con impegno sull'anno successivo, visto che siamo in sessione di bilancio, ritengo che il decreto sia coperto, che siano coperti tutti gli investimenti da assumere per uscire dall'emergenza.

in merito al testo della Commissione, in primo luogo esprimo un apprezzamento per il lavoro svolto, perché questo testo riformulato dopo l'osservazione della Commissione bilancio,

il rischio che addirittura fondi dei campani andassero al Ministero e non al commissario e dall'altro sanciva il principio che i Comuni devono fare mutui. Proprio perché in passato spesso i Comuni sono stati inadempienti, e quindi vi sono dei crediti verso il commissariato sul titolo smaltimento, bene sarebbe stato, come previsto dalla precedente impostazione del relatore, autorizzare i Comuni a contrarre mutui, con un rilievo ovviamente al patto di stabilità. Pertanto, viste le osservazioni della Commissione bilancio e la riformulazione presentata, la mia proposta è di appoggiare così com'è l'emendamento 5.100 (testo 3), verificando se eventualmente in un ordine del giorno si può recuperare la questione dei mutui.

quelli che di fatto hanno portato a un esborso di 80 milioni di euro con il precedente decreto-legge del 2005, prendendosi in più anche i soldi della tassa sui cittadini,

Mi sembrerebbe assurdo pensare di proporre ai cittadini delle altre Regioni una situazione differente, per cui ci sono i Comuni amici degli amici del centro-sinistra che tanto non pagano mai e gli altri Comuni onesti chiamati a pagare tutti i giorni.

che esso, inizialmente presentato dal relatore, prevede un procedimento di immediato accredito al commissario di risorse per i Comuni che non sono riusciti a percepire alcuna somma da parte dei cittadini. I Comuni, in questo caso, si vedono detratto l'importo dal trasferimento erariale e sono così molto più sollecitati, dovendo contrarre dei mutui corrispondenti, ad assolvere ai loro obblighi di riscossione di un'imposta che sappiamo essere evasa quasi al 90 per cento e, quindi, nell'ambito dell'ordinarietà dell'imposta si trovano le risorse. L'approvazione di questo emendamento, tra l'altro - mi rivolgo alla maggioranza e al Governo - integra perfettamente la previsione fatta in sede di approvazione dell'emendamento suggerito dalla Commissione e e sostenuto dal Governo. Quindi è indispensabile per «far cassa» e perché i Comuni vengano responsabilizzati poi nell'attivarsi ad assolvere alla riscossione ordinaria della TARSU.

in parte già richiamata dal relatore e mi pare, in un intervento, dall'onorevole Ronchi. La ritengo abbastanza importante. Questo decreto-legge si incrocia con un altro decreto-legge relativo alle ordinanze che dispongono dell'utilizzazione di risorse finanziarie e si dovrebbe presumere che per tutto il 2006 dovesse essere già coperto finanziariamente dal precedente decreto-legge. Sia chiaro che lo sforzo che noi facciamo è aggiuntivo rispetto a quello che doveva essere ordinariamente previsto dal precedente decreto‑legge e non sarebbe nemmeno giusto non poter mantenere la linea di utilizzazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti percepite in Campania perché quelle sono devolute all'ufficio del commissario delegato, al netto delle somme di ristoro che vanno date ai Comuni nei quali si localizzano gli interventi di raccolta. È evidente che tutto l'insieme della norma finanziaria, così come è stata costruita, ha un suo equilibrio ed è anche evidente che, per quanto riguarda il 2007, bisognerà assicurare la copertura complessiva delle molteplici attività nelle quali il commissario deve

Grazie,

*(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il tema della gestione dei rifiuti, o se si vuole essere più precisi del loro smaltimento, si misura nella capacità del Governo di dare risposte immediate e concrete ai problemi del territorio, a maggior ragione quando si parla della Campania, Regione martoriata dall'emergenza

gli effetti di un approccio sbagliato, dovuto al facile ricorso dello smaltimento finale in discarica come unica via di gestione*.* Al dì la delle legittime osservazioni espresse da numerosi colleghi circa le responsabilità e le colpe dell'attuale condizione, è il momento di guardare oltre. Siamo in una situazione di emergenza massima. Dobbiamo affrontare il problema dei rifiuti nell'ambito della maxi problematica ambientale laddove va programmata una buona politica per venire a capo della complessità della questione. È il momento di rispettare ruoli e gerarchie istituzionali affinché la politica, agendo in un'ottica in un'ottica *super partes*, possa sovrastare gli interessi di pochi ed arginare il fenomeno dell'ecomafia che per troppi anni ha imperversato, mettendo in ginocchio l'intero sistema. Le misure dettate dal decreto-legge - peraltro lacunoso - e modificate opportunamente in Commissione e in quest'Aula rappresentano solo un punto di partenza nelle more del passaggio ad una gestione ordinaria, auspicio di molti. Occorre, infatti, sottolineare lo sforzo compiuto in Commissione ambiente, dove, nonostante il duro scontro e l'iniziale disaccordo, come forza politica abbiamo ottenuto le necessarie modifiche migliorative al testo, come quella relativa alla limitazione del commissariamento in Campania, strumento cui ricorriamo da troppi anni. L'emergenza rifiuti in Campania fu dichiarata nel lontano 1994 ed è ora che di emergenza, dopo questa fase, rientrando nell'ordinario, certamente non si parli più. più. Non possiamo indugiare ancora nel commissariamento, procedura straordinaria, nata come scorciatoia per la soluzione del problema, al contrario totalmente improduttiva. Oltre al termine ultimo di rientro nella gestione ordinaria, si è ottenuta l'espunzione della norma che sanciva l'utilizzazione *ex lege* delle tre discariche individuate dall'articolo 5 del provvedimento. Il sopralluogo effettuato insieme ad altri delegati della Commissione ambiente aveva dimostrato, infatti, che Tufino, così come le altre due discariche, è come un bicchiere colmo d'acqua al quale non si può aggiungere neanche una goccia. Ben più correttamente, allora, la norma modificata dispone che il commissario deve individuare ed utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti siti di stoccaggio e discariche tenendo in debito conto il carico ambientale e i disastri provocati dalle discariche o o da altri impianti esistenti in evidente stato di saturazione. Ora, dobbiamo sostenere serie politiche di intervento per uscire da questo stato critico. Dobbiamo, ad esempio, far capire che i termovalorizzatori ad alta tecnologia e ad impatto ambientale zero sono l'unico rimedio, la risposta razionale alla problematica, nonché una consistente risorsa energetica ed economica. Anche noi, imitando i Paesi più evoluti, dobbiamo intelligentemente trarre energia dai rifiuti, così questi, da fardello dispendioso per i cittadini, diventeranno fonte di risparmio e contemporaneamente avviare quel processo di normalizzazione attraverso l'incentivazione alla raccolta differenziata che da obiettivo elementare, partendo dal singolo cittadino ligio, raggiunga la collettività dando un apporto a tutta la Regione. Viceversa, senza una corretta raccolta diversificata, i cittadini resteranno in ogni caso ostaggio della spazzatura. Voglio dire che i particolari poteri dati a Bertolaso, con la collaborazione di tutte le istituzioni, rappresentano l'*incipit* e devono essere considerati solo il mezzo per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è ripristinare l'ordinario e la regola in Campania. Da ultimo, lodevole è l'iniziativa di cui all'articolo 2 del decreto che oggi stiamo per convertire, che prevede misure volte ad incrementare la partecipazione e l'informazione dei cittadini che vivono ancora nel caos. Da campano, infatti, mi avvilisce dover constatare che gli stessi cittadini esasperati mentre contestano la riapertura delle discariche e fanno barriere impedendo ai camion carichi di sversare, contraddittoriamente poi danno danno fiamme agli enormi cumuli di spazzatura senza riflettere sugli innumerevoli danni ambientali e alla salute provocati da simili gesti. Ecco perché, a nome del Gruppo che rappresento, dichiaro il voto favorevole al provvedimento. È d'uopo più che mai non esitare nella conversione del decreto in oggetto e - delegato dal Capogruppo

Signor Presidente, ci troviamo nuovamente oggi a dover procedere alla conversione di un decreto che il Governo ha emanato sotto la spinta della necessità e dell'urgenza. Questa volta, effettivamente, la situazione a cui si cerca di porre rimedio ha i contorni dell'emergenza, ma amaramente constatiamo nuovamente un'emergenza conosciuta e annunciata. La gravità del problema dei rifiuti si aggiunge come un macigno ai già mille problemi di una Regione martoriata e - purtroppo bisogna anche sottolineare ormai governata da diversi anni, una quindicina, da amministrazioni di sinistra sia alla Regione che al grande Comune di Napoli che non hanno saputo agire in maniera efficiente ed incisiva. É cronaca di questi giorni, infatti, un'altra gravissima emergenza che coinvolge il capoluogo campano, ormai terreno di scontro della criminalità organizzata che miete vittime anche tra la popolazione della città. Anche per questa ulteriore situazione il Governo corre ai ripari con provvedimenti di urgenza senza mai mettere in discussione l'operato della sinistra in quei territori - è una situazione un po' paradossale, poi parlerò anche delle affermazioni di Bassolino in relazione a queste responsabilità -, senza mai predisporre dei provvedimenti realmente incisivi che comportino riforme strutturali per eliminare le cause di tutto ciò. Amaramente di nuovo ci troviamo qui a discutere su un provvedimento frettoloso, mal congegnato e mal meditato. Si tratta di un provvedimento che non riesce a dare ossigeno ad una Regione che muore soffocata tra i fumi dei rifiuti, frutto dell'operato di un Governo che non riesce ancora a dare risposte convincenti, a diversi mesi dal suo insediamento. L'inadeguatezza delle istituzioni a far fronte a situazioni come queste è oggi purtroppo evidente. Oggi i cittadini si sentono meno tutelati e più soli. Napoli, sotto il peso della criminalità, e la Campania tutta sotto quello dei rifiuti, soccombono ignorate dai propri amministratori, colpevoli di politiche scellerate e personalistiche. Il resto dell'Italia, del popolo italiano, assiste indignato, ma noi oggi qui non possiamo rimanere in silenzio, assecondando così coloro che del silenzio e del malcostume hanno fatto una bandiera. Ecco perché diciamo no ai continui provvedimenti tampone e chiediamo, anzi pretendiamo, interventi incisivi, strutturali, che individuino soluzioni rapide e definite per problematiche oramai croniche e incancrenite. È doveroso che il Governo, il quale si fregia di essere stato eletto dai cittadini, indaghi con accuratezza e severità le cause e i responsabili che hanno condotto la Campania a dover essere commissariata. I danni all'ambiente, alla salute e ai cittadini sono enormi e richiedono a gran voce giustizia, ma una giustizia vera, che non si risolva in una mera bolla di sapone per offuscare l'opinione pubblica. Non possiamo più accontentarci del solito scaricabarile tra enti locali e Governo centrale, o tra amministratori ed ex amministratori. Chiediamo che il Governo metta in discussione seriamente e definitivamente l'operato dell'intera classe dirigente e gli stessi esponenti del centro-sinistra, che da decenni operano in Campania, abbandonando i facili proclami e le false promesse. È doveroso che Prodi ammetta che, in quindici anni di centro-sinistra, non sono state messe in campo politiche di sviluppo, ma neanche è stata affrontata una questione elementare e basilare come quella dei rifiuti, portandoci oggi qui a dover fronteggiare un'emergenza che ci scredita anche a livello europeo.

- che qui a Roma il traffico o l'impossibilità di imboccare il raccordo anulare siano colpa del duce. È esattamente la stessa affermazione. Anzi, Pomicino e Gava hanno finalmente espresso qualche giudizio sulle amministrazioni che li hanno succeduti, perché non solo niente è migliorato, ma qualcosa è peggiorato e sicuramente quei luoghi sono in mano alla camorra come non mai. Ancora il popolo italiano non ha potuto udire una sola parola da cui possa desumersi una qualche assunzione di responsabilità e i cittadini campani, costretti a respirare gli odori che esalano dai rifiuti che circondano le loro case le scuole dei loro figli, non hanno potuto vantare il diritto di guardare sul viso dei responsabili alcuna forma di pentimento. Sono più di sette anni che l'emergenza rifiuti in Campania è alla ribalta della cronaca: sette anni di fallimento su tutta la linea, nonostante il commissariamento; sette anni di vorticosi giri di denaro, di cui qualcuno ha approfittato, lucrando sulla pelle della gente comune e alimentando la malavita, che oggi impera tra le strade di Napoli come padrona incontrastata del territorio (altro che passato!), di fronte ad uno Stato assente.

i Comuni sono inadempienti. Si dà, finalmente, un mandato per stilare nuovamente il piano regionale dei rifiuti, che in tutti questi anni di commissariamento non è mai stato modificato; non si è praticamente fatto nulla per la raccolta differenziata: questo è ciò che ha portato alla situazione attuale. Finalmente, si danno anche indicazioni chiare per chiudere - speriamo una volta per tutte - la vicenda dell'appalto FIBE, con gli impianti vetusti,

un decreto - e ne sono stati emanati tanti - sull'emergenza dei rifiuti in Campania: è, quindi, la prima volta che esprimiamo un voto a favore e vogliamo sottolineare con forza che sarà anche l'ultima. Si tratta di uno sforzo

Mi pare che «emergenza», che dovrebbe essere - come dice la parola stessa - una situazione straordinaria, qualcosa di improvviso, non lo è in questo caso. Come i Paesi tropicali hanno la stagione delle grandi piogge, così a Napoli, in Campania abbiamo la stagione delle «scoasse», come diremmo noi in Veneto, la stagione delle immondizie. Infatti potete osservare, anche dalle riprese televisive, che esse sono sempre uguali; non sappiamo a quale anno si riferiscano, però vediamo le strade piene di immondizia. Oggi il Governo ha deciso che tocca al capo della Protezione civile, al dottor Bertolaso, che sembra abbia minacciato delle probabili - o

quando la Regione Campania bandisce una gara per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Alla gara, fra gli altri, partecipano ENEL e Impregilo. L'ENEL viene premiata con un giudizio tecnico di 10 ed un'offerta economica che vale un 7. Invece, Impregilo, che ha un'offerta tecnica di 3

con una tecnologia obsoleta ma a prezzi stracciati. L'allora presidente della Regione campana, Losco, capisce che qualcosa non va e non se la sente di assegnare ufficialmente la gara. Ci pensa però il suo successore, il governatore Bassolino, ad assegnare alla famiglia Romiti le chiavi della gestione rifiuti in Campania, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La Campania è stata trasformata da Impregilo in una gigantesca discarica a cielo aperto: dal luglio 2001, infatti, data in cui è entrato in funzione il primo impianto di produzione del presunto combustibile da rifiuti, oltre quattro milioni di «e-balle», le famose ecoballe, pari a oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti, sono stoccate in aree più o meno vicine ai centri abitati. Mi chiedo se qualcuno ha mai fatto una seria indagine sulle proprietà di queste aree, cioè cioè a chi Impregilo paghi elevati contratti di affitto. Torniamo sull'argomento della Commissione di inchiesta dei rifiuti, che ha lavorato nella scorsa legislatura e ha messo in evidenza e in luce come, tra la composizione del prodotto, degli scarti e dei rifiuti di ingresso non vi sia assolutamente nessuna differenza: sono tutti uguali. Questa, a mio avviso, potrebbe definirsi una truffa. Però, nessuno ne ha parlato. È un silenzio omertoso. Sarebbe anche interessante sapere se è vero quanto si mormora, che cioè fra le aziende che hanno ricevuto regolarmente, nel corso del 2006, dal commissario il pagamento della fattura, ci sia solamente l'Impregilo o anche altre. Così vedete che, mentre l'Impregilo guadagna, i rifiuti restano in strada e il commissario viene spedito su un'altra trincea.

che fino al marzo 2004 è stato lui il commissario sulle cosiddette scoasse, come le chiamiamo nella mia Regione; crede di nascondersi trovando altri capri espiatori. Credo che il governatore Bassolino farebbe meglio a non cercare foglie di fico e ad assumersi le proprie responsabilità. a tutti i cittadini italiani, di qualsiasi Regione, tocca pagare di tasca propria l'esportazione dei rifiuti campani, pagare di tasca propria l'esportazione dei rifiuti campani, è perché in cinque anni, come commissario, Bassolino non è riuscito ad individuare un solo sito per realizzare gli impianti di smaltimento.

si registra la maggiore evasione di tale tributo, e - io aggiungo - anche di altri! Mi chiedo soprattutto come pensa il Governo di sanare gli oltre 400 milioni di euro di debiti accumulati dalle passate gestioni

Poche settimane fa il ministro Pecoraro Scanio ci ha raccontato in Aula magnifiche e progressive sorti proprio per la Campania, visto che il termodistruttore di Acerra è pronto a partire e che altri sono in via di costruzione.

un provvedimento - rischio di sembrare contraddittorio - anche necessario, perché chi conosce i problemi di questo settore, che la Campania vive ormai da troppi anni,

È una situazione difficile quella della Campania, non solo per quanto riguarda il settore dell'emergenza rifiuti. Però voglio ricordare, come ho fatto in sede di discussione generale, che il problema rifiuti è un elemento determinante, che inquina tutta la vita della Campania, anche per quanto riguarda la cosiddetta emergenza criminalità, la cosiddetta emergenza ordine pubblico. Voglio sottolineare che il problema non è di Napoli ma di tutta la Campania. Certo, a Napoli è molto più forte, molto più visibile, molto più duro, però è un problema campano in generale. È un problema che riguarda le discariche; che riguarda il trasferimento di rifiuti tossici che arrivano da tutta Italia: lo voglio ricordare da uomo del Nord (non

C'è una necessità, perché in Campania ci guadagnano tutti tranne che i cittadini. I cittadini continuano a pagare e voglio ricordare, come ho già fatto, specialmente tutti quei cittadini onesti - e sono più di quanto pensiamo che le tasse, forse meno che in altre Regioni del Paese, le pagano e che con questo decreto, che -ripeto - lascia aperti dei margini di discrezionalità, rischiano - speriamo di no - di pagarle

il problema della tariffa, resto convinto che bisognasse scrivere chiaramente in questo provvedimento che la tariffa dei rifiuti non si può aumentare. perché il rischio è che, come accade per le tasse in tutto il Paese, l'elevazione della tariffa la paghino sempre coloro che hanno continuato a pagare senza avere un servizio. Questo provvedimento non chiarisce lascia ampi margini di interpretazione. È per questa ragione che non possiamo esserne completamente soddisfatti. Così come non possiamo essere soddisfatti della parte che riguarda l'individuazione dei siti. Quando si parla di rifiuti (e questo vale spesso in tutto il Paese, specialmente quando ci sono emergenze, perché queste non sono solo quelle fortemente visibili, come quella della Campania, ma ve ne sono in tutto il Paese), quando si tratta di individuare individuare un sito di stoccaggio, i comitati e i cittadini che insorgono si trovano in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta fino a Trapani. Dunque, il problema esiste. Allora, cosa accade spesso? è più comodo utilizzare quei siti che hanno già dato la disponibilità, quei territori dove i cittadini hanno già pagato, elevarne magari la capacità di accoglimento di rifiuti

da altre aree della Regione. Dunque, è evidente che anche qui, anzi ancora più qui che in altre aree nel Paese, chi è virtuoso non ci guadagna assolutamente nulla. Durante Durante le nostre audizioni abbiamo ascoltato i presidenti delle Province, i quali hanno sostenuto tutti, indipendentemente della formazione e dal colore, la necessità di provincializzare. Io continuo a sostenere la necessità di corresponsabilizzare gli enti locali nella soluzione di un problema che è stato creato dalla politica - lo dico chiaramente - e dall'incapacità dalla politica di guidare le scelte.

di chi ha fatto le grandi scelte nella storia d'Italia e nella storia d'Europa. Dunque, io credo che non si debbano fornire alibi

sull'emendamento che aumentava i poteri al commissario sulla gestione delle cave, perché riteniamo che il presidente di questa Regione debba assumersi totalmente le responsabilità politiche ma anche le responsabilità tecniche nel risolvere un problema. Non può scaricare tutto completamente completamente sulle spalle di Bertolaso e del Parlamento che, come ho già detto, in questa sede, pur non avendo colpe, si è impegnato a collaborare insieme a quell'area del Paese, alla Regione, che non ha collaborato. Ripeto: Bassolino non si è degnato nemmeno di venire in audizione! Il Parlamento ha lavorato per risolvere un problema del Paese, giustamente, perché noi dobbiamo essere insieme corresponsabili, perché non vogliamo - lo ripeto - e non conviene a nessuno, anche se qualcuno ogni tanto ci pensa, avere un Paese a due velocità, un Paese di serie A e uno di serie B. Conviene a tutti avere un Paese che cresce velocemente, di pari passo, dunque dobbiamo aiutarci. Voglio ricordare anche al senatore Schifani che la questione della FIBE è stata sollevata fin dall'inizio, fin dall'inizio, anche dal sottoscritto, perché l'anomalia è proprio quella che la FIBE, guarda caso, da quando è stato rescisso il contratto, guadagna molto, molto più di quello che guadagnava prima anche perché tutti i conti le vengono pagati immediatamente e *cash*. Dunque ritengo che non si debbano fare polemiche sui lavori socialmente utili non utilizzati, sui mezzi che vengono pagati e spariscono, ma ho ripetuto questi aspetti solo per un motivo: perché voglio chiamare tutti a un atto di corresponsabilità. In Campania sono necessarie delle regole: il Parlamento ci ha messo buona volontà

che dobbiamo svegliarci e dobbiamo continuare a seguire il Paese, perché dobbiamo da qui guidarlo continuamente. Proprio per i motivi che ho detto, l'UDC si impegna a mettercela tutta per migliorare la situazione in un area del Paese difficile.

che la 13a Commissione è stata impegnata sulla materia sia attraverso un sopralluogo in Campania, sia attraverso audizioni, sia attraverso un pesante lavoro di verifica e modifica del testo. Devo manifestare una notevole perplessità per l'evidente incompiutezza del testo del decreto-legge governativo e soprattutto per le incertezze in tema di copertura finanziaria, come stigmatizzato dalla 5a Commissione nel suo parere, estremamente articolato, del quale la 13a Commissione si è fatta ampiamente carico. Il quadro generale di queste disposizioni fa riferimento, con tutta evidenza, ad una situazione nella quale l'emergenza è ordinarietà, tanto è vero che la materia è stata ripetutamente oggetto di simili interventi legislativi da anni a questa parte. Dalle audizioni, in particolare, è emerso uno stato preoccupante di disarticolazione fra le diverse istanze amministrative locali, Comuni, Province e Regione. Tra l'altro, mi pare umiliante per il Senato della Repubblica, che sta intervenendo per conto di tutti e a carico anche della fiscalità generale, per diminuire una situazione locale di disagio, che il presidente della Regione Campania si sottragga a confronti in sede istituzionale. In taluni momenti è parso, in sede di 13a Commissione, ma anche qui in Aula, di trovarsi anche a dover sostituire gli amministratori locali addirittura nel farsi carico di dettagli, quali le specifiche allocazioni delle discariche. Credo che, se oggi si decide di intervenire ancora una volta in fase di emergenza, occorra anzitutto esprimere apprezzamento per tutte le realtà locali italiane (Regioni, Province e Comuni) che, diversamente, si stanno impegnando a gestire e risolvere in proprio la questione rifiuti, certo con fatica, ma certo altrettanto ivi compresa quella raccolta differenziata che sta dando buoni frutti, ove fortemente spinta dalle amministrazioni locali. Occorre poi prevedere in Campania azioni molto forti, sia in termini amministrativi (con riferimento alla organizzazione di uffici, alla corretta gestione di gare di appalto, alla decisione circa il destino lavorativo di centinaia di addetti), sia in termini di gestione immediata: quindi, non ci sia chi chiude discariche quando il commissario le apre o le riapre; si accelerino oggi le procedur per la realizzazione di termovalorizzatori; si definisca il nuovo piano rifiuti. Intorno alla scelta di rinnovare il commissariamento, occorre una sollecita presa di coscienza ed un adeguato impegno politico locale verso il futuro. *Tempus fugit*: non ritroviamoci fra un anno a rivedere gli stessi temi nelle stesse condizioni, non accontentiamoci di sistemare la questione trovando i fondi per l'immediato, senza contemporaneamente essere capaci di forzare verso una soluzione di sistema. Poiché riteniamo che il disegno di legge di conversione, così come integrato e corretto in questo tormentato *iter* senatoriale, possa avviare questo processo, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà voto favorevole.

e forse dei nuovissimi che ancora devono arrivare, ma ci si è dimenticati quanto sta succedendo da dodici anni in spregio ai cittadini campani e in spregio a tutti i cittadini italiani, con particolare riferimento ai cittadini di quelle Regioni che il problema dei rifiuti l'hanno risolto da soli, lavorandoci alcuni minuti al giorno, alcune mezz'ore al giorno. Mi riferisco a quelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali che hanno evitato, in questi dodici anni, di buttare nel cestino della spazzatura non riciclabile un miliardo di euro, ovvero 2.000 miliardi di lire: 2.000 miliardi per risolvere i problemi di una Regione, una sola Regione su tutto il territorio nazionale. Questo è assolutamente ingiustificabile, come è ingiustificabile che la politica non abbia voluto identificare i responsabili.

provvedimento deve dire semplicemente una cosa: l'emergenza dei rifiuti campani la deve risolvere la Regione Campania e i fondi necessari non devono più essere succhiati dalle tasche di tutti i cittadini attraverso nuove imposte. Signor Presidente, è un problema che va risolto là: i rifiuti se li tengano in Campania, se li smaltiscano loro! Considero la mia una dichiarazione di dissenso integrativo, perché voterò contro

concretezza di atteggiamento e realismo, nella consapevolezza che sia necessaria comunque una risposta ancora in termini emergenziali, ma parimenti convinta che il problema principale sia politico: il superamento definitivo in Campania della logica dei commissariamenti e non soltanto di questo. Ciò riporta necessariamente a un'amara considerazione circa la politica della gestione del territorio, in particolare ad opera della Regione Campania. Il nostro è stato un contributo significativo proprio in questa logica, introducendo proposte emendative che hanno determinato innanzitutto una limitazione temporale della fase del commissariamento, perché non si parlasse di un commissariamento senza limiti di tempo.

che affligge insanabilmente questo provvedimento: l'effettiva mancanza di risorse per il commissario, tali da metterlo in condizioni di poter realmente operare, nel solco di quello che era stato, viceversa, l'atteggiamento ben più fattivo del Governo precedente negli anni 2001-2006. Lo abbiamo fatto, ma abbiamo dovuto prendere atto in quest'Aula della vostra sostanziale incapacità di risolvere una situazione che è tanto emergenziale da imporre interventi adeguati e concreti, perché dall'emergenza (finalmente, dopo dodici anni) si passi a una fase di normalità.

con il quale si invita il Governo a reperire altre risorse oltre quelle modestissime, oltretutto in conto capitale, che dovrebbero garantire non si sa bene cosa, a fronte dell'impegno finanziario del commissariamento verso gli oltre 2.000 lavoratori socialmente utili, ci porta all'amara constatazione che ancora una volta si tenta di scaricare sulle imprese e sui cittadini campani il costo di una drammatica situazione, attraverso il riferimento a un ulteriore e assolutamente indeterminato, impreciso e nebuloso inasprimento fiscale, con un meccanismo di copertura che potremmo definire a copertura eventuale, differita e addirittura a consuntivo.

che avrebbe voluto che votassimo contro questo provvedimento. Il nostro senso di responsabilità e l'attenzione vera che Alleanza Nazionale ha per i problemi reali del Mezzogiorno ci porteranno ad esprimere un voto di astensione, legato però ad un auspicio, che è, al tempo stesso, un preciso monito al Governo. il Governo trovi fondi adeguati e in questo suo ormai traballante e agonizzante cammino abbia la forza almeno di fornire una risposta concreta ad un'autentica, drammatica emergenza, che riguarda non solo i campani, ma tutti noi. noi. Se percorrerà questa strada troverà la nostra collaborazione, mentre, se le cose resteranno così come sono, graverà su questo Governo e su questa maggioranza la responsabilità di un altro fallimento, così pesante da seppellirli sotto un cumulo di insipienza ben più alto di quello dei rifiuti che drammaticamente soffocano la Campania. Per questi motivi il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà.

che ora vengono chiamati termovalorizzatori. Ecco perché nasce l'emergenza rifiuti in Campania. Vi è stata una decisione folle, imposta dalla sinistra, che verteva su una contraddizione in termini:

Le discariche furono chiuse perché bisognava impedire alla camorra di fare affari. In realtà, si sono chiuse le discariche, è sorta l'emergenza rifiuti, ma la camorra ha comunque continuato a

In Campania si è arrivati al punto che smaltire una tonnellata di rifiuti costa 140 euro, mentre nel resto d'Italia ne costa 50.

Finalmente fu potenziato il NOE, cioè il nucleo dei carabinieri che contrasta il sistema criminale per quanto riguarda l'inquinamento ambientale e si prese atto che bisognava intervenire sulle discariche. Dopo dodici anni e dopo aver sperperato 2.000 miliardi, con una gestione commissariale affidata ad un *manager* di indiscusse capacità come il dottor Bertolaso, noi ora riapriamo le discariche tornando al punto di partenza ma avendo bruciato 2.000 miliardi.

Si calcola che ogni cittadino della Campania sarà gravato ogni anno da una tassa sui rifiuti che oscillerà dai 60 ai 70 euro. Quindi, per un famiglia di cinque persone si tratterà di 350 euro,

i due subcommissari Jucci e Alfieri, due ex generali dei carabinieri, riescano a tenere lontani affaristi, camorristi e imbroglioni dall'emergenza rifiuti.

ma la loro posizione e la loro facoltà di disporre è sempre limitata e mai determinante ai fini dell'individuazione delle aree di stoccaggio. Questo sistema che si tenta di rinnovare non offre soluzioni credibili, vere, realistiche sulla scorta di quanto avvenuto in passato anche, e soprattutto, perché da parte della sinistra non vi è stata un'analisi forte e precisa delle responsabilità. Eppure avevamo come base un documento

con fondi che non si sa dove andare a reperire. Se questa è la situazione, il mio voto non può che essere contrario, richiamandomi anche all'ordine del giorno che non ho potuto presentare, ma che faceva riferimento a questa esigenza per il territorio casertano.

con una motivazione che mi permetto di dire sarebbe censurabile in Cassazione perché dalle premesse non sono state tratte le logiche e giuridiche conseguenze.

è vero che l'emergenza inizia nel 1994, però quest'ultima fase ha delle cause specifiche e si rischia di non focalizzare il problema se si fa di tutta l'erba un fascio. Quest'ultima fase di emergenza deriva dal fatto che il ciclo di gestione dei rifiuti della Campania ha avuto un punto di congestione negli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti: sette impianti che ricevevano rifiuti da tutta la Regione per poi doverli destinare al recupero energetico. Poiché gli inceneritori non sono stati costruiti e quello di Acerra è in ritardo, quei sette impianti si sono ingorgati

Si occupa, infatti, di come risolvere il problema delle 5 milioni di tonnellate di rifiuti che, trovandosi in centri di recupero del CDR, fermano tutto il ciclo di smaltimento dei rifiuti.

al recupero attraverso la produzione di CDR ben sapendo, da anni, che questo CDR non aveva sbocco perché gli impianti per bruciarlo non c'erano e che quindi si pagava per produrre combustibile derivato dai rifiuti e stoccarlo nella consapevolezza della mancanza di impianti per gestirlo. Si interrompe questo ciclo e si avvia uno smaltimento di cinque milioni di cosiddette ecoballe.

La seconda carenza del sistema è la raccolta differenziata. La Regione Lombardia, se non avesse il 42 per cento di raccolta differenziata, fra tre mesi sarebbe in emergenza, anche se è dotata di impianti di incenerimento. Fa il 42 per cento di raccolta differenziata e questo consente di non entrare in emergenza. Anche sulla raccolta differenziata questo decreto ha potenziato molto le misure per supportarla e certo poi ci vorrà la collaborazione degli enti locali e l'impegno dei cittadini. Il terzo fattore così concludo - riguarda il completamento degli impianti tecnologici per il recupero energetico. Penso che l'idea di fare due mega inceneritori a distanza di venti chilometri per tutta la Campania era una scelta sbagliata. Se ne sta facendo uno e questo va completato. Bisogna però che anche nelle altre Province il ciclo sia integrato, qui c'è un dibattito, però bisogna che si arrivi ad una decisione non per bruciare tutto - non c'è nessuna Regione, nemmeno in Europa, che brucia tutto -, ma per completare il ciclo di gestione dei rifiuti. Penso che con questo provvedimento si siano poste delle condizioni utili per uscire dalla fase di emergenza. Abbiamo approvato l'idea di dare una data terminale, la fine del 2007, per la gestione commissariale. Penso che questo sia non solo un impegno politico, ma anche un impegno per consentire effettivamente il superamento di questi snodi nella gestione dei rifiuti in Campania e poter davvero tornare a una gestione ordinaria.

perché stiamo discutendo da tre giorni in quest'Aula di una questione che non dovrebbe esistere. Ci si meraviglia poi che il Paese scivoli in tutte le graduatorie mondiali di qualunque tipo. Stiamo parlando da tre giorni al Senato di rifiuti.

Per andare al succo della questione, finirà come l'altra volta: i rifiuti arriveranno nelle Regioni padane, dove invece i cittadini accettano le discariche, accettano gli inceneritori e fanno la raccolta differenziata. Quindi, per concludere, quando si parla di questione settentrionale - parliamo anche di queste cose - questo è l'esempio di come in Italia le cose non funzionano, ma soprattutto di come si continuano a non farle funzionare, invece che intervenire penalmente